Grazie.

ordini del giorno G 9.106

«assumere una iniziativa legislativa urgente volta a» siano sostituite dalle seguenti: «valutare la possibilita, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in armonia con la generale disciplina generale in tema di assunzioni, di

«La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere precedentemente espresso, formula un parere di semplice contrarieta` sugli emendamenti 11.69, 11.71, 11.225 e 11.226».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 9 agosto. Nella seduta pomeridiana di oggi, il cui orario di chiusura estato posticipato alle ore 20,30, proseguira la discussione del decreto-legge in materia di rilancio dell’occupazione e IVA. Il calendario di questa settimana prevede inoltre l’esame del decretolegge cosiddetto Ilva di Taranto e del decreto-legge in materia di ecobonus, quest’ultimo giaapprovata dal Senato e in corso di modifica da parte della Camera dei deputati. In relazione all’imminente scadenza di tali provvedimenti, gli orari delle sedute sono stati prolungati ed e stata prevista, in luogo del sindacato ispettivo, una seduta con votazioni nella giornata di venerdı2 agosto, nella quale si procedera inoltre, come giastabilito dalla Camera dei deputati, alla votazione per l’elezione di due componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria. La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di lunedı 5 agosto, saranno discussi il decreto-legge in materia di rilancio dell’economia, nonche´ ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri ed eventuali altri decreti-legge giaapprovati dal Senato, ove modificati dalla Camera dei deputati. Il calendario potra eventualmente essere integrato con lo svolgimento dell’interpellanza n. 42, Nugnes ed altri, sollecitata dal presidente Morra. Per quanto riguarda le richieste di votazione nominale con procedimento elettronico, saradata applicazione al parere reso dalla Giunta per il Regolamento il 14 settembre 1992, la quale ha stabilito che: «La richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti. Non vale una richiesta formulata una tantum con l’intento di avere effetto per tutta la seduta». Secondo quanto convenuto dalla Conferenza dei Capigruppo, per gruppi di voti si intende il complesso di emendamenti e ordini del giorno relativi ad un articolo. Infine, non saranno piu ammessi interventi per dichiarazione di rettifica, ritardo o mancata effettuazione di voto, che potranno tuttavia essere comunicati per iscritto ai senatori Segretari (Applausi ai fini dell’inserimento nel Resoconto della seduta, ferma restando l’impossibilita` di modificare il risultato della votazione elettronica di riferimento.

mira ad espungere dal testo della legge una disposizione che prevede che, laddove il contratto collettivo abbia escluso la responsabilitasolidale dell’appaltante la responsabilitasolidale dell’appaltante per la retribuzione del dipendente dell’appaltatore, resta in vita una corresponsabilita dell’appaltante per i contributi previdenziali. si mantenga la responsabilitaper la contribuzione quando invece viene meno per disposizione collettiva la responsabilita per la retribuzione del lavoratore. Poiche´ si tratta di una anomalia, io chiedevo, e torno a chiedere, che il Governo e i relatori esprimano un parere non negativo. Chiedo quale ragione possa mai esservi per creare una diversa disciplina per retribuzione da una parte e contribuzione previdenziale dall«altra.

contrapporre un’osservazione a quella fatta dal collega Ichino. La salvaguardia della responsabilita` solidale sulla quota contributiva ha l’evidente ragione di proteggere almeno la quota dei contributi previdenziali dei lavoratori che incorrono in questa fattispecie allo scopo di preservarne le pensioni. Quindi, noi non siamo favorevoli alla proposta del senatore Ichino.

senatore Ichino.

egarantito dall’automatismo delle prestazioni previdenziali. Quindi, prendo atto della volonta di non tener conto di un’obiezione ragionevole. Avverto pero` che in questo modo si introduce nel nostro ordinamento una norma che a me pare davvero irragionevole.

9.14 vi e un invito a ritirare l’emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno. Chiedo alla senatrice Fuksia se e` d’accordo.

di sostenere le spese per lo svolgimento di attivitasociali anche mediante forme di lavoro accessorio. Questo, a nostro avviso, toglie tanta attivita a quelle cooperative sociali che lavorano sul territorio nel sociale.

La ringrazio

da quelli che sono assoggettati a riduzione in caso di mancata adozione da parte della Regione di misure di riduzione dei costi della politica,

con l’emendamento 10.0.200 si intende ampliare la capacita` delle casse previdenziali con riferimento ai giovani professionisti e alle barriere che essi incontrano nell’accedere alla professione. Fermi restando i saldi di finanza pubblica, nell’ambito di economie aggiuntive a quelle che sono richieste alle stesse casse previdenziali, deve essere possibile lo svolgimento di funzioni di sostegno ai giovani professionisti, come qui si dispone. Mi auguro che il Governo – eventualmente anche suggerendo opportune correzioni – possa accogliere questo emendamento.

Se vuole, rileggiamo il parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992: «La richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti. voti. Non vale una richiesta formulata una tantum con l’intento di avere effetto per tutta la seduta». Lei l’ha fatto sul primo e il senatore Carraro l’ha fatto sull’altro gruppo.

e poi puntualmente ritirati, perche´ tutti i decreti sono assolutamente blindati. C’el’impossibilita di poter interagire con le altre forze politiche e poter votare delle cose di buonsenso. Stiamo assistendo ad una farsa.

parlamentare, eassolutamente evidente che, quando si fa una proposta, compete alla responsabilita dei senatori nell’interlocuzione con l’Aula e il Governo trovare le coperture. Questo emendamento non ha copertura. Pertanto, ho provveduto a ritirarlo e il Governo ha accettato di occuparsi dei contenuti di questo emendamento accogliendo un ordine del giorno, che egia stato approvato. Dal punto di vista procedurale non ho potuto dichiarare ritirato e trasformato in ordine del giorno questo emendamento perche´ un ordine del giorno sullo stesso contenuto estato approvato con riferimento ad un precedente articolo e quindi risulta gia fra gli impegni del Governo.

Il Governo propone la riformulazione

del Regolamento, gli emendamenti 11.12, 11.214, 11.219, 11.220, 11.80, 11.81, 11.235, 11.236

destinati alla Regione Siciliana: tra l’altro esiste a tal proposito un’apposita convenzione tra la Regione Siciliana e il Ministero dell’economia

a patto peroche si rimoduli la somma prevista, per un importo non superiore a 10 milioni di euro.

pagare alcuni rilevanti debiti da parte delle Regioni a statuto speciale con un mutuo pluriennale dello Stato. Per le Regioni a statuto speciale e stata chiesta un’ulteriore garanzia, perche´ lo Stato evidentemente non si fida della loro capacitadi rimborso del mutuo pluriennale.

sulle spalle dei cittadini. Nulla fa la Regione per ridurre le sue spese, ma in realta non fa altro che aumentare il carico fiscale nei confronti dei cittadini. in questi giorni c’estato, a seguito di un articolo di stampa, un balletto di notizie provenienti dalla Regione siciliana. Il Presidente della Regione ha detto che questo aumento non s’ha da fare, l’assessore al bilancio ha detto che e giaconcordato con lo Stato e poi il Presidente e abbiamo una rassegna stampa che in cinque giorni fa cambiare opinione cinque volte agli esponenti del governo regionale siciliano. Detto questo, echiaro che e giastato fatto in sede di presentazione del decreto, quindi un mese fa, un accordo preciso

tassa e di questo aumento dell’imposta regionale siano tali da arrivare sino al punto di coprire ben 30 anni (perche´ qui parliamo di un mutuo trentennale). Ho dunque chiesto se non si potesse ridurre questo importo o se non si potesse limitarlo nel tempo. ministro Fassina mi ha detto che mi avrebbe risposto e spero che lo fara in questa sede. Comunque, io mantengo certamente

la` dove si vincola «esclusivamente» a questo fine l’eventuale aumento dell’imposta regionale. Purtroppo, siamo abituati nel tempo a concedere aumenti, anche

di sapere se puo essere ridotto, come io propongo, nei limiti dello 0,73 piuttosto che dell’1 per cento e, temporalmente, nell’arco di due anni piuttosto che non nell’arco di 30 anni. Sono cifre sulle quali io non ho la disponibilitadei

alla spesa pubblica regionale, sempre che il Governo accetti il cambio di garanzia dall’imposta

Signora Presidente, preannuncio la presentazione di un testo 2 dell’emendamento che, sostanzialmente, tiene conto delle riserve avanzate in sede di discussione generale. L’emendamento riguarda il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e

al pagamento di questi debiti, assistendoli con la garanzia dello Stato e prevedendo l’intervento di enti intermediari finanziari, come gia prevede la legge recentemente approvata. In questo senso chiediamo che l’emendamento venga accolto.

Presidente, intervengo per illustrare l’emendamento

questa decisione come un atto di fiducia. Sono convinto che vi sarada parte del Governo, che desidererei consapevolezza della necessita di porre rimedio ad un problema che resta irrisolto da molto tempo. Nel 1994 con la legge n. 29 il legislatore intese introdurre alcune disposizioni finalizzate a disciplinare la figura del terapista della riabilitazione non vedente, al fine di determinare, tra l’altro, dei benefici sotto il profilo occupazionale. Lodevole l’iniziativa e la premura che il legislatore ebbe all’epoca rivolgendo attenzione ad una platea di soggetti diversamente abili. Cosa eaccaduto? E[ ]accaduto che nel corso del tempo, in particolare negli anni successivi, con l’introduzione della legge n. 42 del 1999 prima legge n. 251 del 2000, sono state introdotte alcune modifiche che hanno comportato l’eliminazione della figura professionale del fisioterapista dal novero delle professioni ausiliarie della sanita. Cio ha determinato, evidentemente, l’impossibilitaper la legge del 1994 di trovare applicazione a beneficio dei non vedenti per un fatto di vuoto normativo e di modifica della terminologia della qualifica di questi operatori. L’emendamento da me presentato era finalizzato a ripristinare una regolarita, ad aggiornare la la tipologia dell’attivitadi fisioterapista e a consentire l’applicazione dei benefici per agevolare l’occupazione dei fisioterapisti non vedenti. Mi e stato chiesto dai relatori l’impegno di trasformare l’emendamento in ordine del giorno. Ho accolto questa richiesta e ringrazio i relatori. Confermo il mio ordine del giorno e lo sottopongo

l’emendamento 11.218, il problema investe l’attivitadei call center che hanno attuato, entro le scadenze previste, misure di stabilizzazione dei collaboratori

di misure di credito d’imposta per spalmare su un periodo piu lungo alcuni benefici, di questa tipologia di imprese eche, a fronte di meccanismi che agevolano ora le nuove assunzioni, rischiano di ritrovarsi completamente fuori mercato essendo la loro attivita per l’80-90 per cento costituita dal costo del lavoro. Mi sembrava fosse un buon proposito rendere durature delle buone misure introdotte qualche anno fa che hanno prodotto stabilizzazione.

sappiamo che esiste un tavolo di confronto con il sistema delle organizzazioni ed il sistema dei gestori delle concessioni a fini turistico-ricreativi,

vorrei spiegare. Vi sono situazioni nelle quali i manufatti amovibili, previsti esplicitamente nel progetto di concessione,

per smontare e poi migliaia di euro per rimontare le strutture. Si tratta di collegare l’insistenza delle strutture per il periodo esclusivo della concessione. Pertanto la riformulazione sarebbe

(…), mantengono installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. Dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

11.0.3. Chiedo pero al Ministro competente di chiarire definitivamente il problema delle sanzioni per le

Attendiamo il nuovo parere della 5ª

abbiamo ritirato i nostri emendamenti relativi al settore dello spettacolo e della ricerca sulla base dell’impegno del Governo ad accogliere un ordine del giorno, che oltretutto eformulato in modo molto

Come ho avuto modo di accennare anche in Commissione bilancio nella giornata di ieri, la previsione contenuta nella norma norma finalizzata alla costruzione di un piano di rientro sugli anticipi che lo Stato da per il pagamento dei debiti alle imprese non ha una particolare caratteristica per le Regioni a statuto speciale. Ciascuna Regione deve far fronte con le proprie risorse al piano ventennale di rientro degli anticipi che prende dal bilancio dello Stato, per saldare i 40 miliardi di debiti che complessivamente Stato, Regioni ed enti locali hanno nei confronti delle imprese, e pertanto si predispongono

in esame euna possibilita per l’amministrazione regionale e la dimensione dell’aumento e` coerente con le risorse necessarie al piano di rientro.

inequivocabilmente solo per questo fine, e diversamente non venga attuato. Chiedo quindi di rivedere il parere solo sull’emendamento 11.209 e ritiro gli altri emendamenti.

il vice ministro Fassina ha appena dichiarato di volere accogliere, aggiungiamo le firme dei componenti del Gruppo PdL della Commissione bilancio. Vorrei ricordare al Vice Ministro, come abbiamo avuto occasione di fare durante i lavori della Commissione di ieri, che

commerciali delle nostre pubbliche amministrazioni: sono quelli che il Governo ha deciso di stanziare per coprire una delle misure piusignificative per la crescita del nostro Paese). L’effetto indotto dal testo che il senatore Santini ha ha predisposto, invece, aiutera e favoriranon solo la rapida esecuzione di tutto questo, ma anche un effetto finanziario positivo, in modo da allargare questa possibilita e quindi immettere nelle imprese preziosa in questo momento, e nel futuro poterne aggiungere altra. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione

volevo dichiarare il mio voto favorevole all’emendamento 11.2, che abbiamo sottoscritto, anche perche´ ha una motivazione.

provvedimento. Sappiamo che sono buoni i dati di trasferimento delle dotazioni finanziarie disponibili al fine del pagamento dei debiti delle

Quei famosi 7,6 milioni di euro che vengono sottratti, in realta vengono sottratti dal fondo per il funzionamento ordinario dell’universita, cioe un fondo che dovrebbe essere destinato esclusivamente a delle voci specifiche. Per questo, eun gioco degli specchi e delle tre carte

a causa di questo emendamento, visto che euomo d’onore, a doversi dimettere. In realta, quel fondo edestinato soltanto alla ricerca, agli stipendi, ai magazzini, alle strutture e alle spese del personale. Quindi, certamente vi e una distrazione di somme destinate ad altro.

l’organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte con

Presidente, lei sa quello che io sto per domandarle: lei ritiene che questa sia una riformulazione o in realtaun nuovo emendamento del Governo? Questo e un nuovo emendamento del Governo, e quindi noi le chiediamo di avere a disposizione il

perche´ questa ela prima volta che si fa uno sforzo vero nei confronti del lavoro nel settore turistico e della cultura nel nostro Paese. Quindi, e un piccolo passo avanti.

Grazie. Vorrei ricordare che si tratta di una modifica utile e tuttavia non tale da risolvere tutte le esigenze del turismo, dei pubblici esercizi e del terziario in generale.

un lavoro subordinato, spesso a tempo indeterminato e con tutele complessive, ma di cui non e ponderabile il momento nel quale effettivamente si avvia la prestazione. Quindi, e` un lavoro che corrisponde spesso imprevedibili, che si manifestano nel lavoro terziario e, in modo particolare, in quello di carattere turistico. Bene quindi abbiamo fatto a rimuovere un Grazie.

Grazie.

il rappresentante del Governo perche´ questo suo emendamento assume lo spirito dell’ordine del giorno legato all’emendamento 7.16, che avevo presentato in precedenza,

la tipologia di rapporto sia per quanto riguarda i soggetti destinatari del provvedimento, eevidente che si tratta di una riformulazione, e non gia di un nuovo emendamento del Governo. Ed e` questa la risposta che va data

Signor Presidente, essendo stato riformulato l’emendamento, va presentata una relazione tecnica conseguente.

Il Governo ha suggerito una riformulazione che e stata accolta dai proponenti e che ha ricevuto l’approvazione e la firma di altri senatori e altri Gruppi politici. che si tratti di una riformulazione in senso sostanziale, e quindi procedo alla votazione.

Mi perdoni per questo mio breve ma irrituale intervento che non riguarda direttamente i lavori dell’Aula. Vorrei solo sottoporre alla sua attenzione l’esigenza (lo ritengo doveroso) di assicurare il rispetto della legge anche – e soprattutto, direi – all’interno dei palazzi della politica. In particolare, mi riferisco alla normativa che regolamenta il fumo sui luoghi di lavoro. Non edifatti ammissibile che i fumatori comuni, all’interno dei comuni luoghi di lavoro, debbano sottoporsi a disagi non indifferenti pur di assicurare il doveroso rispetto della salute di chi non fuma, mentre al Senato della Repubblica si possa tranquillamente fumare, senza che nessuno si preoccupi dell’enorme danno che cio provoca a chi ecostretto a subirne la vicinanza. Non credo sia necessaria una particolare competenza per rendersi conto dell’imbarazzante, costante violazione del divieto di legge, legata vicinanza. Non credo sia necessaria una particolare competenza per rendersi conto dell’imbarazzante, costante violazione del divieto di legge, legata anche alla almeno apparente inadeguatezza dei locali allo stato a cio destinati qui a palazzo Madama. Il rischio ovviamente, oltre al danno personale alla salute che subisce quotidianamente chi – come il sottoscritto – non tollera fisicamente il fumo, equello ulteriore di far apparire all’esterno che la classe politica anche per il fumo goda di privilegi che i cittadini comuni non hanno, il tutto ovviamente nel piu assoluto disprezzo del diritto alla salute costituzionalmente tutelato. Per queste brevi considerazioni, signor Presidente, confidando nel suo amore per la legalita, mi permetto di invitarla, per quanto di sua competenza, ad attivarsi per la realizzazione anche all’interno di questo prestigioso palazzo di un’adeguata e regolare area dedicata a chi purtroppo non intende o non e ancora riuscito a liberarsi dal vizio

Prego i colleghi di allontanarsi dall’Aula in silenzio, per favore, per consentire gli interventi.

Il Parlamento eappassionato ormai da tempo ad un dibattito direi rilevante per gli assetti democratici del Paese, che si riferisce in particolar modo all’architettura dello Stato, al superamento del bicameralismo paritario, al migliore rapporto fra potere esecutivo e legislativo,

Dobbiamo fare veramente molta strada, in questa pur collaudata democrazia, per vedere riconosciuta la dignita di chi svolge questa funzione, signor Presidente. Con rammarico, devo dirle che sono costretto paradossalmente, dopo ben otto richieste scritte rivolte al Ministero dell’istruzione

che fa parte di una procedura in atto fra il Ministero dell’istruzione e il TAR del Lazio.

della borsa di studio agli specializzandi. Io chiedo l’acquisizione di un documento che il magistrato amministrativo ha chiesto al Ministero di produrre nell’ambito di un contenzioso. L’ho chiesto da oltre un anno a questa parte; non ho avuto riscontro; sono stato costretto ad avanzare un’interrogazione parlamentare nello scorso mese di aprile

portano talvolta a percorrere le strade secondarie e non i viali e a chinare il capo, chissaper dover scontare quali gravissime colpe. Signor Presidente, io adempio al mio dovere con umilta e anche con diligenza e tenacia e ritengo che si possa fare di piue meglio nel Paese per salvaguardare la democrazia e servire il popolo. Finanche, signor Presidente, la dignita di questo Parlamento e quella di questo ramo del Parlamento potrebbe anche trovare un miglior riscontro nel trattamento che viene riservato ai senatori in tante occasioni. Abbiamo rinunziato anche al ristorante, perche´ era opulento nell’offerta ed economicamente troppo oneroso; per carita,

emortificante ed umiliante, se si considera che anche la breve sosta di due minuti per guardare la televisione, per leggere i giornali e mantenersi informati sui fatti del territorio, che prima

gli uffici hanno giasollecitato piu volte la sua interrogazione, l’ultima volta – mi dicono – addirittura di recente, fino a qualche giorno fa. Speriamo di poter ottenere l’effetto desiderato.

un intervento a difesa del Senato della Repubblica e dell’attivita` che ciascuno di noi svolge. Noi in Commissione giustizia abbiamo lavorato in questi mesi e, come lei sa, durante la seduta della settimana scorsa quando c’era il Ministro della giustizia, ho ricordato in quest’Aula che abbiamo ritardato per tre mesi l’approvazione in Commissione giustizia di una proroga della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in quanto il Ministro ha chiesto incontri con la maggioranza parlamentare al fine di verificare possibilita` di apportare correttivi. Signor Presidente, Presidente, dopo che la Commissione giustizia ha votato all’unanimita`, stamattina senatori del PD, del Movimento 5 Stelle e del PdL hanno chiesto la calendarizzazione

e i Presidenti delle due Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno dimostrato al Ministro la disponibilita anche a una proroga di soli tre mesi e a individuare i correttivi necessari. Ci sono cittadini che non hanno nessun mezzo di collegamento con il tribunale a cui sono stati aggregati, e parlo di aree industriali del nostro Paese vicino Milano. E allora, signor Presidente, come Presidente del Senato, mi rivolgo a lei perche´ intervenga nella riunione dei Capigruppo affinche´ questo Parlamento e quest’Aula abbia la possibilita` di discutere

il Governo ha detto che ein atto un lavoro per cercare di trovare soluzioni equilibrate. Siccome lei mi invitava a parlarne nella riunione dei Capigruppo, la informo la risposta del rappresentante del Governo e, quindi, io aspetterei ulteriori risposte. Proprio il presidente Morra aveva presentato questa una cosa che non fosse la realta! Non c’e nessun rapporto da piudi venti giorni! Quindi, non mi venga a dire una cosa che non e reale. Non mi sarei mai permesso di offenderla riferendole una cosa non reale. ma di cosa stiamo parlando? Ho detto che la sua stessa richiesta e` stata presentata nella riunione dei Capigruppo.

con parole cosıpesanti figure importanti, che lavorano al servizio dello Stato da molti anni, credo che la Presidenza debba prendere in considerazione la possibilita di intervenire. Naturalmente non pretendo di aver ragione, ma ho ritenuto giusto segnalarle il caso. Esprimo altresı, a nome mio e del Partito Democratico, la totale e assoluta vicinanza alla procura di Torino, al procuratore Caselli e ai procuratori Rinaudo e Padalino, che stanno esclusivamente svolgendo il loro lavoro, che e quello di applicare la legge.

All’epoca fu individuato perche´ in quel sito gia erano contenute scorie provenienti dagli Stati Uniti d’America ed erano barre di uranio che servivano per alcune sperimentazioni di arricchimento di uranio utili al nostro Paese. All’epoca si disse che prima o poi quelle barre d’uranio sarebbero dovute rientrare negli Stati Uniti d’America. Lunedıscorso, alle 3 del mattino, ingenti Corpi di polizia hanno provveduto a spostare quelle barre d’uranio e a riconsegnarle,

una violazione delle prerogative del Parlamento, e del Senato in particolare, il fatto che non sia stato calendarizzato subito un provvedimento che estato votato all’unanimita in Commissione giustizia. Ricordo che la calendarizzazione urgente estata richiesta praticamente da tutti i Gruppi. Il Governo ha posto una questione di mero temporeggiamento, cosa che sta facendo da mesi:

sono ore di ansia per la sorte di un padre gesuita, padre Paolo Dall’Oglio, di cui si sono perse le notizie poche ore fa mentre era nel Nord della Siria.

dove solo poche ore fa ci sono state 106 vittime accertate in un attacco alla cittadi Homs, di cui 13 bambini e sei donne. Sono solo le ultime vittime di una guerra civile che, secondo le Nazioni Unite, ha gia causato causato 100.000 morti. Credo che si tratti di una vicenda drammatica che avviene quasi alle porte di casa, in questo piccolo laghetto che si chiama mar Mediterraneo, nel quale conviviamo con altri Paesi, e che purtroppo si svolge un po’ nell’indifferenza generale. Soprattutto, si svolge nella totale assenza di una politica da parte dell’Europa e dei suoi alleati, anche americani. Sostanzialmente, di questo Paese nessuno si sta veramente occupando e nessuno ha un’idea di che cosa si debba fare. Credo che l’Italia, per il ruolo che ha sempre rivendicato all’interno del Mediterraneo, debba porsi con un atteggiamento di maggiore responsabilita. Ritengo che si debba aprire un dibattito

cercando in questo modo di interpretare al meglio la missione di questo padre gesuita, il quale ha consacrato la sua vita al dialogo interreligioso, a portare

verra in Parlamento e mi auguro che voglia cogliere questa opportunita` per raccontare e spiegarci quali sono le iniziative che il Governo intende promuovere in questo senso. (Applausi